recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, premesso che: l'articolo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

agli eventi meteorologici estremi che si sono verificati a partire dalla giornata di domenica e si sono protratti in gran parte del territorio lombardo e piemontese, rivelandosi particolarmente violenti e preoccupanti nella provincia di Como

colpita la riva occidentale, nel Comune di Blevio, dove sono state evacuate persone. I filmati che abbiamo potuto vedere

territorio è molto fragile, di una bellezza incredibile, ma, proprio per tale ragione, le rive così scoscese e i corsi d'acqua e i torrenti che scendono al lago rendono la situazione difficilissima, quando cade una pioggia intensissima in così poco tempo. Il terreno bagnato non riesce a drenare e si formano quelle cascate di fango che tutto portano al lago.

da Cernobbio e Tavernola fino a Colonno; tutti i torrenti si sono ingrossati e le immagini sono davvero spaventose. Il panico ha preso le persone, che hanno visto portare via le macchine;

sono state sospese le forniture d'acqua in alcuni Comuni, ma soprattutto sono stati molto colpiti Moltrasio, Laglio, Argegno, Colonno e Cernobbio,

necessaria la dichiarazione dello stato di emergenza, perché i danni sono veramente molto ingenti. Gli abitanti del lago di Como, i cosiddetti laghee, sono persone molto schive e lavoratori ma hanno subito un colpo incredibile alle loro case e hanno paura per la salute e per l'incolumità delle proprie famiglie. È un territorio prezioso, non solo per la provincia di Como, ma per l'intera Italia, perché è uno dei luoghi turistici più belli, più affascinanti e più apprezzati dai turisti stranieri. Spero ci sia molta attenzione non solo da parte della Regione Lombardia, ma anche del Governo tutto. un grido di dolore: salviamo e proteggiamo il nostro territorio. Anche se le piogge erano previste, davanti a una simile quantità di acqua e alla violenza della grandine e del vento, poco si è potuto fare.

di una zona fondamentale anche sotto il profilo economico, quindi è giusto che le venga dato rilievo e che ci sia la vicinanza di tutto il Paese a una popolazione tanto colpita. ringrazio, senatrice Rivolta. Naturalmente, a nome dell'Assemblea, esprimiamo solidarietà alle famiglie, alle amministrazioni locali operatori economici, le cui attività sono state colpite da questa calamità. Sicuramente non mancherà l'attenzione del Parlamento per i provvedimenti necessari, che purtroppo sono sempre più frequenti a causa delle emergenze climatiche.

recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

per consentire la trattazione degli argomenti in esame, le vorrei chiedere di poter intervenire a fine seduta per illustrare le richieste che provengono dalla Sardegna a seguito della dichiarazione

e perché alla Camera è stato al centro di un dibattito ricco e articolato, fino a restituirci un testo indubbiamente migliorato. Penso in particolare all'allargamento del tavolo permanente con i rappresentanti della cittadinanza attiva e all'inclusione nella cabina di regia dei rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane. Penso alle migliorie apportate rispetto al controllo e alla verifica dei processi e anche ad alcune modifiche di merito, come quella che amplia il bonus del 110 per cento per scopi di utilità sociale, quali ospedali e case di cura. Tutto questo è l'ennesima conferma dell'importanza dell'attività parlamentare e della centralità che le Camere devono avere su provvedimenti così importanti. lo dico anche con un po' di invidia per i colleghi della Camera e con rammarico poiché, sullo strumento che stabilisce le regole per i prossimi anni, qui in Senato ci limitiamo a un passaggio meramente burocratico; ed è un peccato, perché permane ancora una serie di nodi da sciogliere. Mi riferisco in particolare alla partecipazione delle autonomie speciali a tutti i finanziamenti del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari Questa deve avvenire indipendentemente dall'estensione delle tipologie di competenza che caratterizza le singole autonomie e delle relative responsabilità nel loro finanziamento. Inoltre, dando per scontato che le risorse del *recovery* non sono riconducibili alla fiscalità generale nazionale, la partecipazione delle autonomie a questi finanziamenti dovrà prescindere da eventuali regole e meccanismi finanziari e contabili che regolamentano i rapporti finanziari tra Stato centrale e autonomie speciali. Allo stesso tempo, nella cornice dei vincoli e degli obiettivi del PNRR, va salvaguardato il ruolo di regia e di coordinamento che le autonomie speciali svolgono rispetto ai Comuni, in ragione della competenza in materia di finanza locale. Se tutto questo non avvenisse, sarebbe semplicemente assurdo e potrebbe costituire materia per contenziosi e ritardi nell'uso delle risorse. Ci auguriamo che Governo e singoli Ministeri si attivino sulle risorse del PNRR e del PNC di propria competenza per definire criteri adeguati di accesso alle risorse o di modificare quelli attualmente applicati

il rallentamento delle vaccinazioni, i dubbi e le proteste sul *green pass*, nonché le scelte da compiere per una riapertura ordinata dell'anno scolastico. Come ho detto la scorsa settimana, l'unità nazionale si dimostra anche sostenendo scelte che nell'immediato possono risultare impopolari, ma che alla lunga fanno crescere la credibilità dello Stato e la fiducia verso le istituzioni. Per questo, non voglio neppure immaginare quanta sfiducia verso il sistema Paese si verrebbe a determinare se l'Italia non riuscisse a spendere gli aiuti europei. Bisogna continuare a lavorare per la semplificazione, per sciogliere i nodi che ancora permangono sulla gestione delle risorse, per le riforme strutturali, *in primis* la giustizia, e per sviluppare progetti credibili e utili alla crescita dei territori, motivo per cui è di vitale importanza il protagonismo anche degli enti locali. Non dobbiamo solo fare in fretta; dobbiamo anche fare bene. Questo provvedimento è il pilastro attorno al quale si possono fare entrambe le cose. Per questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie.

all'effettiva digitalizzazione del Paese, con il pieno coinvolgimento dei giovani in un settore che è nelle loro corde, e a raccogliere effettivamente la sfida che abbiamo davanti, attraverso le disposizioni di inclusione, per promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere, l'assunzione dei giovani

inoltre preziose misure di semplificazione delle procedure di appalto e qui è d'obbligo il richiamo al decreto-legge semplificazioni del 2020, con cui abbiamo permesso l'accelerazione delle procedure, con deroghe importanti al codice degli appalti. Per una migliore applicazione, però, sarebbero forse serviti degli accorgimenti in più, ma sottolineo anche che abbiamo bisogno di una classe dirigente in grado di applicare regolamenti e leggi con competenza, per un vero sblocco della burocrazia, che spesso non è dovuta solo al coacervo di norme, ma anche alla negligenza e all'incapacità di agire a tutela degli interessi dei cittadini e del settore pubblico o privato. In questa direzione va anche la previsione che, da un lato, conferisce la realizzazione operativa degli interventi previsti alle amministrazioni centrali, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti locali, sulla base delle loro specifiche competenze e attraverso le proprie strutture, dall'altro, determina un potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza da parte di uno dei soggetti attuatori, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR. Si tratta di un'assunzione di responsabilità da parte dello Stato non di poco conto, che però necessariamente deve far scaturire altrettanta responsabilità nei soggetti attuatori, che devono agire con professionalità, utilizzando gli strumenti per realizzare gli investimenti pubblici e con un chiaro aumento di efficienza di ogni attività. Rilevante è poi la disposizione che prevede l'applicazione delle misure e delle procedure di velocizzazione anche ai progetti contenuti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, estendendo le procedure finanziarie alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, i cui 15,5 miliardi del PNRR, si interviene in modo incisivo sulla struttura tecnica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, creando un procedimento *ad hoc* per una serie predeterminata di opere di particolare rilevanza strategica, interamente finanziate, che devono realizzarsi rispettando il cronoprogramma prefissato. Tra queste, mi permetto di ricordare la realizzazione dell'asse ferroviario Palermo-Catania-Messina

con agevolazione estesa all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti e con possibilità di fruizione oltre il 2022, non essendovi un limite temporale all'utilizzo in compensazione. Come referente nazionale di Italia Viva per le aree interne sono soddisfatta anche delle norme che, intervenendo sulla strategia nazionale, consentiranno di attuare gli interventi individuati con la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati e il coordinamento del Ministero per il Sud e la coesione territoriale. anche l'accelerazione per le procedure relative ai beni confiscati alle mafie, per il tempestivo svolgimento delle attività sugli interventi di valorizzazione di questi beni, con possibilità, per quelli non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica, di essere utilizzati dagli enti territoriali, oltre che per le finalità di lucro con reimpiego dei relativi proventi, per finalità sociali, anche per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria. Colleghi, da parlamentare del Sud ho notato particolare attenzione e varie misure a favore del Mezzogiorno nel decreto-legge all'ordine del giorno. Ora mi rivolgo ai territori del Sud, a chi li rappresenta nei vari livelli amministrativi e politici. Il Meridione può essere veramente protagonista per le grandi potenzialità da cui può partire lo sviluppo, promuovendo il Sud, anziché denigrando sempre il lavoro fatto, evidenziando strumentali differenze. Le risorse ci sono dico ai colleghi parlamentari, ma anche a chi mi ascolta dai territori, che, piuttosto che piangersi addosso, devono essere bene investite per realizzare quanto si può e quanto si deve ai cittadini, senza stare a contare gli spiccioli in più o in meno rispetto alle altre Regioni. L'Italia è una e, finché non lavoriamo e pensiamo in un'ottica anche visionaria di Paese-Italia in un contesto europeo e internazionale, difficilmente ci libereremo da pregiudizi e dall'annosa questione meridionale, tirata in ballo con rimpianto da parte di alcuni nostalgici dei tempi borbonici, utilizzando impropriamente il richiamo alla Magna Grecia, che ancora è lì davanti ai nostri occhi, assuefatti da una nebbia che ci fa essere miopi, senza renderci conto che le opportunità sono a portata di mano. Una di queste, forse la più importante per unire veramente il Paese e per rilanciare il Mezzogiorno, creando migliaia di posti di lavoro e assicurando un riscatto morale e sociale per i nostri giovani e le imprese, è la possibilità concreta di realizzare il ponte sullo stretto di Messina. Non è più una leggenda, ma un sogno che si avvera, grazie a tre fattori in sinergia mai verificatisi prima: il fronte politico favorevole sempre più ampio, di cui prova l'intergruppo parlamentare che mi onoro di aver promosso; la grande determinazione dell'ingegner Pietro Salini, pronto a sostenere in gran parte l'opera con Webuild; e la piena disponibilità delle Regioni Calabria e Sicilia di rivolgersi al mercato finanziario per reperire i fondi mancanti. Un Governo che punta sulla crescita non può che essere a favore di quest'opera e ringrazio il presidente Draghi che sta seguendo direttamente il *dossier* e ha dato disponibilità di incontrare appena possibile una delegazione dell'intergruppo. Con questo Governo c'è veramente spazio per una nuova visione e per dimostrare una capacità che va oltre, al di là di bandierine politiche e di discorsi, per ridare fiducia alla nostra meravigliosa Italia, facendoci riscoprire, con l'umiltà dei grandi, la dignità di essere donne e uomini dello Stato. Per queste ragioni, annuncio il voto favorevole del

poter essere stanco per i lavori della Commissione; magari vorrei aver trascorso la nottata ad esaminare emendamenti e ad apportare modifiche a un importante decreto-legge che potrebbe essere essenziale e basilare per la realizzazione del PNRR. Vorrei tanto essere qui oggi magari a svolgere un intervento non sulla fiducia, ma sul merito

brutta via, intrapresa ormai da troppo tempo. Ne abbiamo parlato più volte, io stesso ne ho parlato la scorsa settimana:

se nelle prossime settimane continuerete imperterriti con questa violazione delle norme costituzionali e a non accogliere i richiami del Presidente della Repubblica. Non vorrei poi ricordare - ma lo faccio ugualmente, perché credo sia utile soprattutto per il Governo - quello che ho detto la scorsa settimana, cioè che il 95 per cento dei decreti attuativi previsti dal Governo Draghi è ancora non realizzato. Questo vuol dire che la potenzialità delle normative e degli interventi dello Stato di fatto viene limitata quasi integralmente,

minimamente incidere su un provvedimento, e ad esprimere ormai un voto quasi rituale di fiducia al Governo, da parte peraltro, cari colleghi, della maggioranza forse più ampia della storia repubblicana, dall'estrema sinistra ai nostri alleati di centrodestra, gli amici della Lega e di Forza Italia. Siete tutti insieme, avete la più grande maggioranza e, nonostante ciò, ricorrente al voto di fiducia.

come da sempre fa, di migliorare con qualche proposta e con qualche progettualità i decreti che arrivano nelle Aule parlamentari. Nonostante tutto questo, ricorrete continuamente al voto di fiducia. i cittadini lo devono sapere - che ricorrete al voto di fiducia per scappare dai problemi intestini che caratterizzano la vostra maggioranza, che politicamente di fatto non esiste e quindi regge un Governo al quale è demandata quasi la totale autonomia nel decidere le sorti del Paese. Avete affidato il Paese a un Governo che è libero, nei fatti, di fare quello che vuole, quindi le Camere hanno rinunciato al ruolo che la Costituzione e le regole democratiche imporrebbero Il Senato poi - mi auguro che la presidente Casellati voglia far sentire al più presto la sua voce - ormai da qualche mese emarginato dai principali provvedimenti del Paese, che vengono approvati e discussi alla Camera e arrivano qui per una semplice passerella. Ringrazio quindi il presidente D'Alfonso per aver accolto l'appello che Fratelli d'Italia, anche per mio tramite, ha rivolto la scorsa settimana, chiedendo a tutti i rappresentanti istituzionali, ai Presidenti delle Commissioni *in primis*, di rivolgersi ai Presidenti delle Camere affinché insieme, nella tutela della democrazia e della Costituzione, si rivolgano al Presidente della Repubblica. Il presidente D'Alfonso ha accolto questo richiamo. So che ha scritto una lettera

la strada per un più facile approdo dei fondi in economia e un più facile ribaltamento dei benefici finanziari nel tessuto economico del Paese. C'è bisogno di semplificazioni e tanta necessità

che fuoriescano dalla normativa specifica ed entrino in quella ordinaria. Abbiamo bisogno di semplificazioni ovunque e non solamente nell'attuazione del PNRR. Questo è un passaggio che dobbiamo capire ed estendere a tutte le nostre realtà normative nazionali. Penso agli appalti, alla sanità, alle infrastrutture e a tutte quelle barriere all'entrata che impediscono da anni, purtroppo, che i capitali nazionali e internazionali affluiscano nel nostro Paese proprio a causa di queste difficoltà, che vanno eliminate. allora, non si è colto questo decreto come occasione per andare oltre, non solo facendo il necessario compitino sul PNRR, ma estendendo il progetto di semplificazione all'intera normativa e all'intero tessuto giuridico su cui si svolgono le attività e i progetti normativi? Signor Presidente, c'è il tema della burocrazia, un altro aspetto che

Arcuri sta tornando di nuovo a essere un beniamino della maggioranza politica. Signori, qui chi davvero viene emarginato è la politica e a non essere più considerate sono le Istituzioni democratiche. Purtroppo veniamo governati da personaggi - ne ho citati due, ma ce ne sarebbero molti altri che non hanno alcuna investitura popolare e che invece, purtroppo, determinano le sorti del nostro Paese. Signor Presidente, concludo con qualche

Provvedimenti che di per sé sarebbero anche positivi e che andrebbero estesi a tutte le Regioni italiane che lo volessero, non devono entrare nelle partite all'interno della maggioranza, con una mancia a qualcuno, piuttosto che a qualcun altro.

(sul digitale, sul 5G, sul *cloud*), ma le contraddizioni della maggioranza non lo hanno permesso. La chiusura nella fiducia non ci permette di dare un

dal finanziamento del PNRR e del Next generation EU non possa essere sprecata. C'è piena consapevolezza tra le forze politiche, soprattutto di maggioranza a giudicare dall'ultimo intervento, del fatto che questi finanziamenti andranno spesi presto e bene - non c'è alternativa al riguardo - con una precisazione in più: non ci saranno alibi, perché c'è una misurabilità chiara di quel che avverrà.

nei prossimi anni rispetto al 2019, l'Italia ce l'avrà fatta, la politica ce l'avrà fatta e il rilancio dell'economia sarà un fatto concreto. E, quando un obiettivo è misurabile, tutti sono maggiormente tenuti ad impegnarsi affinché questa misurazione porti ad un giudizio assolutamente positivo. Il decreto in esame è

di approccio a determinate spese. Il decreto affronta infatti praticamente tutti i temi che vanno trattati. Si parte dall'organizzazione della gestione delle risorse, dalla *governance*, dal monitoraggio del Parlamento e farò un inciso su questo tra poco. Affronta poi i temi della valutazione di impatto ambientale e della valutazione strategica ambientale, non solo per fortuna per le opere del PNRR, ma giustamente anche per quelle

degli incentivi, ma soprattutto delle regole per gli investimenti in fonti rinnovabili, del superbonus: anche qui, con qualche miglioramento intervenuto durante l'esame alla Camera, non c'è proroga, ma snellimento delle procedure della sola CILA. Si affronta il tema della digitalizzazione e poi, con grande precisione, si interviene in alcuni punti degli appalti, quindi della realizzazione delle opere pubbliche, che sarà la parte su cui farò un *focus* maggiore nel mio intervento. intervento. Per quanto i temi siano diversi e disparati, mi pare di vedere chiaramente un disegno organico, una cifra, che è quella cui facevo riferimento prima, che contraddistingue tutti i diversi interventi. In poche parole potrei dire che si lavora per fare presto e bene, con efficienza e con trasparenza, con attenzione per l'ambiente, ma contro le idee di blocchi ingiustificati e indiscriminati rispetto a investimenti necessari decisamente migliorato il testo e qui non posso che unirmi alle riflessioni fatte da altri colleghi: è chiaro che c'è un rimpianto per non averlo potuto fare anche noi. Avevamo anche noi in Commissione cose da dire, misure da mettere in campo. Non è stato possibile: si capisce la gravità del momento, si capisce che bisogna correre e corriamo, rinunciando, ahimè, a un ruolo che ci sarebbe piaciuto svolgere come Partito Democratico in questo ramo del Parlamento. I miglioramenti della Camera sono anche nella direzione di un maggior coinvolgimento del Parlamento, che potrà giudicare semestralmente ciò che sta accadendo. Sul ruolo di Comuni e Province, oltre che Regioni, nella cabina di regia c'è un fatto importantissimo (io dico per noi parlamentari del Sud, ma è facile dire che lo sia per l'Italia),

per garantire anche che in tutti gli organismi di *governance* ci sia la parità di genere: anche questo mi pare un fatto positivo. Sugli appalti il Governo si è comportato esattamente come aveva annunziato. Quando abbiamo approvato le risoluzioni in materia di PNRR, sugli appalti il Governo avrebbe agito in due modi differenti: tutto quello che era urgente sarebbe stato oggetto di un decreto-legge, quello che stiamo discutendo, mentre si rinviava ad una legge delega una revisione più complessiva e generale del codice degli appalti. Ciò è avvenuto, perché la legge delega è stata presentata e assegnata al Senato e all'8a Commissione,

la programmazione, la progettazione e l'acquisizione di pareri, che è sempre il punto più delicato; interviene poi sugli affidamenti di servizi e di lavori, l'esecuzione, il collaudo e le controversie. Nella maggior parte dei casi vi è un rafforzamento e un differimento di data di alcune previsioni che già nel decreto-legge semplificazioni, approvato nel mese di settembre dello scorso anno, avevamo messo in campo con il precedente Governo. che avevamo ritenuto potessero rimanere in vigore solo fino a dicembre 2021 (anzi, nel testo del decreto c'era scritto giugno), sono portate giustamente e pragmaticamente al giugno 2023, perché è di tanto tempo che abbiamo bisogno e probabilmente anche un po' di più. Ad esempio, è potenziato e il collegio tecnico-consultivo, uno strumento molto importante per evitare controversie, così come il salvacondotto per la responsabilità erariale. Già col precedente Governo ritenemmo di dare un segnale importantissimo ai funzionari della pubblica amministrazione: si sentano protetti nel caso di eventuali errori fatti in buona fede, ma si sentano non protetti in caso di omissioni. In sostanza, è un modo per cercare di superare il tema della paura della firma. È stato prorogato anche l'appalto integrato: questa è una misura su cui il PD ha dato il consenso con un po' di sofferenza, avendo sempre ritenuto che la centralità del progetto esecutivo fosse alla base

qualche dissapore, ma si sappia, per esempio, che la Salerno-Reggio Calabria, la Taranto-Potenza-Battipaglia e la Genova-Ventimiglia oggi sono a quel livello di progettazione e se le si vuole realizzare entro il 2026, non c'era altra scelta.

e una soprintendenza centralizzata rispetto a queste opere. Quest'ultima per me è una misura importantissima, perché troppe volte vediamo sul territorio nazionale una difformità nei pareri delle soprintendenze, che è di per sé una discrezionalità elevata, che rende diverse le diverse zone del Paese. Speriamo che funzioni, perché è una scommessa importante. Altri punti saranno affrontati nella legge-delega: uno tra tutti è la qualificazione e la riduzione delle stazioni appaltanti. Qualche volta un po' provocatoriamente mi capita di dire che un ottimo codice con una pessima stazione appaltante non farà realizzare le non farà realizzare le opere, mentre un'ottima stazione appaltante, anche con leggi non buone, arriva alla realizzazione dell'opera. Quindi quello è uno dei temi fondamentali, ma ne parleremo quando arriveremo alla legge delega. Dicevo si tratta di una grande scommessa che dobbiamo vincere e dobbiamo farlo insieme. C'è una parola bellissima nella mia cultura politica che è "sussidiarietà": bene, questo è un caso in cui politica, pubblica amministrazione, funzionari e imprese debbono ciascuno fare la propria parte e nessuno la parte degli altri. Questo approccio virtuoso ci farà vincere la scommessa. Siamo un grande Paese, dobbiamo affrontare i prossimi mesi ed anni con spirito positivo ed entusiasmo, consapevoli che ci si chiede una cosa difficile e fondamentale:

purtroppo, per l'ennesima volta negli ultimi tempi, a dover arrivare a licenziare un provvedimento senza poterlo non dico

a un vero e proprio strappo. Lo voglio dire perché riguarda evidentemente anche il ruolo di questa Camera

in una situazione in cui bisogna certamente correre, ma credo che stia nella responsabilità di quest'Assemblea, e anche dei Capigruppo, trovare un modo perché tutto questo non possa più accadere, perché viene meno il ruolo: qui si sta

qualcuno ha avuto la possibilità di dire qualcosa in discussione generale. Il provvedimento non ha avuto i pareri anche delle Commissioni che erano direttamente coinvolte; l'ha avuto, in realtà, ma praticamente senza esaminarlo. Penso alla Commissione ambiente e anche alla Commissione lavori pubblici, che hanno competenze molto rilevanti sui

del provvedimento. Penso che noi abbiamo una grande responsabilità; una responsabilità che è di tutto il Paese e quindi, a maggior ragione, dei decisori politici.

della messa a terra dei progetti, ma non si possono di nuovo recuperare modelli, anche di semplificazione, che nel passato sono stati fallimentari. Faccio alcuni esempi per essere molto chiara.

e un modello chiaro presenti in tutte le accelerazioni e in tutte le procedure di semplificazione. Guardate, noi dobbiamo sapere che il Next generation EU

perché noi riusciremo a rimettere il nostro Paese nelle condizioni non dico di partenza, ma anche di andare molto oltre e di vincere la nostra scommessa se coinvolgeremo i cittadini. Il PNRR deve essere un modo anche per far partecipare pienamente e coinvolgere i cittadini.

dovrebbe essere quello il nostro articolo 81! Ogni opera dovrebbe essere esaminata da quel punto di vista. Questa sarebbe la grande rivoluzione. *(Applausi)*. Noi avevamo le competenze e la possibilità

È assolutamente incomprensibile come si possa pensare di rendere più spedite e rapide le procedure, mantenendo l'infrastruttura e una burocrazia barocca e ottocentesca, così come, in effetti, si è voluto fino a questo momento. Ringraziamo il Signore che adesso c'è Mario Draghi, presidente del Consiglio dei ministri, che la pensa diversamente dal

onorevole Deborah Bergamini, che qui è in rappresentanza del Ministero per i rapporti con il Parlamento. Siamo tutti consapevoli

abbiamo per non aver potuto contribuire nel merito, nemmeno in minima parte, nemmeno in termini di discussione in Commissione, come lei ben sa,

mi rendo conto che è assolutamente necessario, ma colgo l'occasione per ribadire, ancora una volta, che c'è assoluta necessità di una riforma. Non è più possibile continuare a rimanere inerti di fronte a una situazione rispetto alla quale - ormai sono passati più

davvero ne usciamo fuori male. il provvedimento interviene per la seconda volta, a distanza di pochi anni, su un tema, che è quello dell'approccio barocco, ottocentesco, della nostra burocrazia che agisce anche dietro l'illusione della trasparenza, dell'impossibilità, secondo alcuni, di intervenire contro la corruzione se non attraverso una serie di impedimenti infrastrutturali, di

a una rapida successione di eventi riguardanti la nostra pubblica amministrazione, quindi, la realizzazione di opere e in sintesi di risposte ai cittadini. Il

il Governo Conte 2 abbiamo cercato di intervenire in modo molto più efficace. Personalmente ho prodotto decine di emendamenti per sbloccare la situazione degli appalti pubblici

ringraziando il Signore, c'è un Governo che invece si è reso conto che bisognava andare oltre quel tipo di ostruzionismo, quella visione ottocentesca superatissima, che altri Paesi hanno superato da tempo, che

rende più difficile l'intervento della corruzione. Cari colleghi, è l'esatto contrario: la semplicità è sinonimo di onestà e correttezza, perché laddove c'è semplicità è difficile ci

Con la semplicità no. Qui si viene incontro anche a questo tipo di soluzione; è un altro passo avanti, ma non certo l'obiettivo finale: il codice degli appalti resta quello che è, però, siamo comunque soddisfatti dei passi in avanti che sono stati compiuti, che sono conseguenza del ruolo che l'Italia, con questo Governo, sta cominciando nuovamente a riconquistare. Il Governo Draghi ha prodotto anzitutto il Piano di ripresa e resilienza, un primo obiettivo fondamentale che ha dato la possibilità di chiedere all'Europa una serie di aiuti agli investimenti che si traducono in circa 200 miliardi di euro, che danno un'opportunità vera al nostro Paese di rilanciare la propria economia dopo un anno di depressione e di crisi economica terribile. Ebbene, bisogna saper cogliere quest'occasione. Tutti noi conosciamo i problemi storici che il nostro Paese ha avuto, soprattutto nelle Regioni del Sud; anche quando potevamo attivare

di burocrati che lo hanno consentito. E non è solo colpa della politica, o magari lo è anche, per l'amor di Dio. Una cosa è certa, allo stato attuale abbiamo

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza necessita quindi di procedure più snelle, più rapide, più veloci e di maggiore fiducia verso la politica e gli e gli amministrativi. Questa è la verità, questo bisognava fare e questo si sta cercando di fare con il secondo decreto semplificazioni. Il Governo sta riconquistando uno *standing* e un'autorevolezza che aveva perduto in Europa e l'Europa sta conquistando un posizione che, evidentemente, prima non aveva. La crescita

Senato. Dobbiamo dunque ringraziarli per l'opera che stanno svolgendo e per il passo in avanti che si sta portando avanti. Pertanto, diciamo con fiducia che

un provvedimento importante, quasi uno spartiacque e quindi inizialmente non posso che evidenziare un piccolo problema,

Oggi invece, fortunatamente, andiamo verso un nuovo metodo, che è quello della Lega di Governo, che punta sullo sviluppo del Paese e sulla creazione di lavoro.

Veniamo da un passato in cui è stata resa palese la nostra vulnerabilità e andiamo incontro a un futuro di incertezza alla qualità della vita. Adesso abbiamo un'occasione e per questo oggi è ancora più importante avere successo in quello che facciamo. Quante volte la politica ci ha provato? Sarà questa la volta buona? Se ci riusciremo, se tutto il Paese assieme ci riuscirà, allora vorrà dire che saremo riusciti a superare una fase di stagnazione che dura da troppo tempo e questo per colpa della burocrazia, per colpa La Lega oggi è al Governo per questo,

Per questi motivi noi siamo al Governo e vogliamo restarci. Abbiamo subito costanti tentativi di escluderci dall'Esecutivo; c'è un evidente asse a Sinistra, che tra l'altro è sinonimo di egoismo a discapito del volere degli italiani, perché è abbastanza ovvia questa miopia politica che va a minare l'unità dell'azione del Governo, infastidendo anche il presidente Draghi e creando divisioni totalmente

Qualcuno forse rimpiange il PNRR di Conte, quello che l'Europa stava per bocciare. Sappiate però che questo non funziona, perché la Lega sta qui, determinata, un baluardo per la difesa degli italiani. *(Applausi)*. Noi siamo il primo partito perché il Centrodestra è maggioranza nel Paese e perché vogliamo che i soldi servano agli italiani. Dobbiamo lasciare un'impronta nel presente per riuscire a impostare in maniera proficua il futuro; dobbiamo impostare un metodo del fare e del fare bene; dobbiamo abbandonare gli sprechi e l'improduttività; dobbiamo pensare a cosa serve veramente oggi, abbandonare un'ideologia assolutamente fuorviante e malata e basarci sulla concretezza. Usciamo da un periodo molto buio per la società,

Oggi dobbiamo rilanciare il PIL, dobbiamo iniziare una nuova ricostruzione, abbiamo l'occasione per impostare un nuovo sistema di lavoro che sia efficiente e con un metodo proficuo. Dobbiamo produrre lavoro e abbandonare l'assistenzialismo. Gli italiani vogliono i fatti. È giusto quindi lavorare sui temi che impattano sulla vita degli italiani in modo positivo e che creano benessere; è sbagliato, dall'altra parte, perdere tempo su leggi insensate e, come dicevo prima, ideologiche. A me non interessa, ad esempio, sapere se si mettono insieme due uomini o se si mettono insieme due donne, a me interessa che le persone riescano a mettere insieme un pranzo con la cena, perché oggi fuori di qui non è così. *(Applausi)*. A me interessa che un papà possa fare un regalo a suo figlio a Natale, a me interessa che una mamma possa guardare il suo bimbo pensando che ha un futuro; non mi interessa assolutamente che

Abbiamo quindi inserito nel provvedimento temi seri e impattanti per lo Stato, abbiamo cercato di individuare con chiarezza chi fa cosa, abbiamo dato la possibilità di nominare commissari per sveltire le pratiche, abbiamo individuato abbiamo individuato delle priorità, abbiamo fornito i mezzi per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, abbiamo lavorato a favore delle imprese, inserendo semplificazioni che fossero reali, rendendo possibili delle accelerazioni procedurali, abbattendo quindi alcuni impedimenti burocratici; abbiamo lavorato per i cittadini. Un esempio su tutti è il super bonus per l'edilizia, o una nuova gestione dell'ambiente, dell'impatto e del dissesto idrogeologico. Stiamo finalmente facendo la cosa giusta, perché si è perso troppo tempo. Le persone hanno perso fiducia nella politica; in effetti come si può dar loro torto, quando c'è una parte dell'Emiciclo che tratta le partite IVA come se fossero, a prescindere, dei delinquenti? Non dimentico che qualcuno in questa sede ha chiamato gli imprenditori "prenditori" e questa sarà per sempre la vostra vergogna, sappiatelo. Noi non siamo fatti così, così, ci fidiamo degli italiani e pensiamo che ci sia solamente bisogno di lasciarli lavorare. Crediamo che non ci sia bisogno di uno Stato opprimente, ma di uno Stato che sia a fianco degli italiani. *(Applausi)*. che ci sia bisogno di un nuovo patto di fiducia con gli italiani, perché se non diamo fiducia non possiamo pretendere che gli italiani diano fiducia al Parlamento. Termino, Presidente, da dove avevo iniziato, cioè sottolineando che questo è un provvedimento veramente importante, uno spartiacque che ha la nostra fiducia, perché è privo di ideologie e di propositi insensati; è

*(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è passato giusto un anno da quel luglio del 2020, quando Giuseppe Conte riuscì a rivelarsi perno centrale nell'estenuante trattativa che portò all'accordo tra i *leader* del vecchio continente sul Next generation EU. Di quel periodo ricordiamo la diffidenza che si respirava in quest'Aula, ricordiamo i titoli di scherno dei principali quotidiani nazionali. Adesso c'è uno sforzo trasversale per cercare di dimenticare l'importanza di quel passaggio. Adesso si dice un'altra cosa, ovvero che che il PNRR è un'opportunità irripetibile per il nostro Paese, si usa la classica metafora del treno che passa una sola volta, un treno sul quale il Paese deve assolutamente salire. Diciamo

neanche un centesimo deve andare sprecato, ma quei 230 miliardi devono fare dell'Italia un Paese verde, un Paese che sia modello di rispetto

piangiamo. Abbiamo infatti perso il valore di cosa significa rispettare la terra. Il provvedimento che ci apprestiamo a convertire servirà quindi a definire il quadro normativo nazionale per agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR.

va segnalato: lo hanno fatto i colleghi del MoVimento 5 Stelle durante la discussione generale e devo ribadirlo anche io. Così come per il cosiddetto decreto sostegni-*bis*, parliamo di provvedimenti di importanza capitale per il futuro dell'Italia, nei quali sono scritti il presente e il futuro dei nostri figli, delle nostre imprese e della nostra società e non possiamo ridurre il Parlamento a

Le decisioni della politica devono essere più condivise possibili se vogliamo superare le riserve mentali e le paure dei nostri concittadini. Il MoVimento 5 Stelle ha un capitale di idee, principi e valori che vuole portare in dote al Paese e spendere. Dobbiamo anzitutto ribaltare la convinzione che parlare di ambiente significhi mettere un freno alla crescita e all'iniziativa economica: questa è la prima missione che dobbiamo perseguire.

L'efficientamento energetico e il miglioramento antisismico degli edifici privati non sono più cose da visionari, utopisti e sognatori. Oggi, mentre noi parliamo da questi scranni, i cantieri già avviati con il nostro superbonus del 110 per cento sono prossimi a quota 30.000. I cantieri sono stati aperti per un valore pari a 4 miliardi di euro. Tutto questo è avvenuto grazie al cocciuto lavoro dei miei colleghi del MoVimento 5 Stelle,

sono un traguardo raggiunto procedendo a marce ridotte. Il superbonus (perdonatemi il paragone e la metafora ippica)

è fondamentale che questo possa avvenire attraverso un prolungamento senza distinguo fino a tutto il 2023 e i benefici in termini di ricadute economiche e occupazionali sono giganteschi.

La necessità di spendere nei prossimi anni velocemente non ci deve assolutamente far retrocedere rispetto alla sicurezza del nostro territorio, alla tutela ambientale, ai presidi di controllo e monitoraggio degli interventi pubblici. Mettere a terra risorse nel nostro Paese in modo rapido e sicuro è possibile,

- non solo torneremo indietro, ma torneremo indietro di trent'anni, lo abbiamo detto, e falliremo purtroppo le missioni che ci siamo dati, sia quella della transizione ecologica, sia quella della semplificazione per il miglioramento dei tempi. A maggio Tomaso Montanari scriveva nella rubrica «Emergenza cultura» su «Il Fatto Quotidiano» che la semplificazione di Draghi equivale ad abbattere il freno delle regole, citando il responsabile commercio e lavoro di Forza Italia, che aveva dichiarato che tra le vittime del Mottarone

uccise le regole. Non c'è più un'ideologia che ci sostiene e questo è grave. Abbiamo solo un'ideologia trionfante, quella che demonizza le regole.

massimo ribasso e il subappalto libero, poi frenato dai sindacati, nonostante le centinaia di morti anche durante il *lockdown* sui luoghi di lavoro. dominanti è difficile resistere, perché l'unica regola che bisogna togliere è sempre quella della corresponsabilità; semplificare e tagliare: questa bandiera deve avere le mani libere. Si costruiscono quindi Ministeri, procedure speciali, commissariamenti, silenzi-assensi per aggirare le regole. Da Berlusconi allo sblocca Italia di Renzi La invito a concludere, senatrice Nugnes. Ai colleghi che rumoreggiano vorrei evitare di doverli richiamare uno per uno.

ambientalista tra virgolette, proposta dal Governo, scatena le trivellazioni, resuscita gli inceneritori con il CIP6, il nucleare e apre le porte al CSS libero e al ponte sullo Stretto. Questo è il futuro che ci aspetta. Signor Presidente, l'Alternativa c'è voterà contro questa ennesima fiducia al Governo e contro l'ennesimo schiacciamento autoritario delle prerogative parlamentari. Ormai il ruolo del Parlamento risulta totalmente esautorato: è avvalsa la prassi di esaminare i decreti-legge in sede di conversione in una sola Camera, con l'altra chiamata solo a ratificare. Stiamo votando, come ormai di consueto, l'ennesimo decreto *omnibus*, nonostante i recenti richiami anche del Quirinale. Ci aspettavamo una diversa reazione su questo modo di procedere, soprattutto da parte dei nostri ex colleghi, che nella scorsa legislatura avrebbero fatto le barricate, sia contro il contenuto di un decreto simile che soprattutto contro l'imposizione continua e praticamente scontata della questione di fiducia. Pensate: ben sette voti di fiducia in meno di cinque mesi con il governo Draghi. Il decreto semplificazioni è un provvedimento poi a dir poco *omnibus*: contiene norme eterogenee e variegate, che nel corso dell'*iter* alla Camera è stato letteralmente infarcito dei contenuti più stravaganti. Alla Camera poi è successo di tutto: il lavoro continuamente rinviato in notturna, in modo da non permettere di capire cosa accadesse realmente. Qui al Senato poi è stato umiliante e vergognoso: il testo è stato fatto approdare a due giorni dalla scadenza definitiva. Quanto al contenuto, purtroppo, c'è ben poco da dire: si dà un calcio ben assestato al codice degli appalti, favorendo meccanismi collusivi e clientelari. Si ipoteca la gestione del PNRR, istituendo una cabina di regia *ad hoc*, creando un inutile e costoso mostro burocratico. Si sventra il codice dell'ambiente con nuove norme in materia di VIA e VAS, senza tener presente la tutela del territorio. C'è poi l'aumento degli affidamenti diretti e il ritorno all'appalto integrato: quindi meno controlli e maggiore facilità nell'aggirare le regole. Si tratta di una visione distruttiva del Paese, dove prevale l'autoritarismo delle scelte e noi siamo contro questa visione, contro le *lobby*, contro la logica del "liberi tutti", senza dibattito democratico. I nostri colleghi alla Camera di Alternativa c'è hanno provato a cambiare queste norme e non ci sono riusciti. Al Senato non è stato proprio permesso, ma il problema è rappresentato da chi oggi vota a favore di questo provvedimento e, conseguentemente, di questo Governo: ce lo saremmo aspettati da tutti, tranne che tre anni fa parlava di fare qualcosa di assolutamente diverso dai partiti tradizionali, per cui i principi erano l'ambiente e la trasparenza, ma di questi principi non è rimasto più niente. Concludo, ribadendo convintamente il no di Alternativa c'è a questo Governo e a questo provvedimento. Signor Presidente, colleghi, non darò la fiducia a questo Governo e voterò contro questo provvedimento. Per motivare il mio voto contrario farò solo un piccolo elenco di criticità relative al provvedimento che conta ben 120 articoli: un decreto-legge che riduce ulteriormente la partecipazione del pubblico ai procedimenti per la realizzazione delle opere del PNIEC e del PNRR. Chiuderemo ancora la bocca ai cittadini e le pubbliche amministrazioni che faranno questo costringeranno il pubblico a parlare davanti all'autorità giurisdizionale. Questo provvedimento elimina completamente i criteri per l'individuazione delle aree idonee alla costruzione di impianti di energia. di energia. Si conoscono solo per grandi linee le opere, ma non ci sono più vincoli, perché sono stati eliminati e c'erano nel decreto-legge semplificazioni dell'anno scorso. Tra i molteplici emendamenti che ho proposto c'è proprio quello per rivedere e reintrodurre i criteri a favore della tutela degli ecosistemi naturali e del nostro patrimonio culturale. Si introducono poteri sostitutivi particolarmente invasivi e corsie preferenziali per la VIA e per la valutazione di impatto sulla parte culturale: un'invasione di campo sulla competenza delle istituzioni. Si mette ancora mano alla disciplina sulla posidonia, un paradosso tutto italiano: si stanziano 400 milioni nel PNRR a tutela degli ecosistemi marini, ma poi andiamo a distruggere la posidonia, quindi la costa, che produce il pescato di pregio italiano. Ma dove vogliamo andare? La mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. Nel Cilento ho denunciato con un esposto la difformità che sta portando la gestione sbagliata di tale

la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2332, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,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

Vincenzo,

anche a pagare un tributo in termini di vite umane, com'è capitato in passato. Questa volta fortunatamente non ci sono state vittime tra la popolazione, che però adesso è davvero in ginocchio.

anche quelli selvatici, bruciati o asfissiati dal fumo. La situazione, tra l'altro, non è ancora definita, perché alcuni focolai ogni tanto riprendono vigore non si può non osservare che fatti del genere capitano sempre quando ci sono giornate particolarmente ventose, il che la dice lunga sul fatto che si tratti evidentemente di incendi dolosi: si è accertato che almeno due su tre sono frutto della mano umana.

però, abbiamo bisogno ancora una volta di atti concreti, di interventi urgenti. C'è bisogno di consentire a chi è rimasto senza nulla, a chi ha perduto una vita di lavoro di ripartire, rimettersi in moto e riprendere una vita normale, cosa che sarà estremamente difficile, se è vero com'è vero che, solo per il reimpianto delle piante andate perdute e incendiate, ci vorranno almeno venti anni. È necessario che ci si muova. È necessario che il Governo faccia sentire, al di là delle parole che - ripeto - sono state immediatamente portate all'attenzione di noi sardi,

fatto gravissimo, possa riprendere in maniera adeguata. Quindi, l'auspicio è che il Governo intervenga immediatamente, anche con misure provvisorie, e poi si vedrà strada facendo come agire, eventualmente prevedendo ulteriori misure successivamente, anche nella prossima legge di bilancio. Grazie, Signor Presidente, anch'io voglio approfittare di questa occasione per recuperare davanti ai nostri occhi le immagini devastanti delle fiamme che in Sardegna divorano ettari di macchia mediterranea e minacciano pericolosamente alcuni centri abitati. Ma voglio anche recuperare - ahimè le immagini del mio Salento, che da mesi è violentato da fenomeni che investono ettari ed ettari di pineta storica, nel più vasto comprensorio turistico di Otranto, andati in fumo nei giorni scorsi. Allo stesso modo, da mesi centinaia di ulivi secolari, già seccati dalla xylella, sono diventati il terribile combustibile per incendi facilitati anche dall'afa, che è conseguenza dei cambiamenti climatici. Con il PNRR noi ci siamo impegnati, come Parlamento tutto, abbiamo assunto la responsabilità di costruire un sistema Paese migliore da lasciare in eredità ai nostri figli, investendo in particolare sulla transizione ambientale e quindi anche sul verde. È per questo che ho voluto fare questo intervento: certamente per esprimere vicinanza a chi è stato vittima di episodi del genere - molte famiglie si sono trovate a combattere con queste vicende

per ogni albero secco vittima degli incendi, di impegnarsi con un nuovo albero verde e giovane. Abbiamo questa responsabilità e credo che tutto il Parlamento possa impegnarsi ad esprimere e a concretizzare una relativa Signor Presidente, una delle zone più incontaminate dell'isola di Sardegna, una lingua di territorio che parte dai pendii del Montiferru, contrassegnati da fittissimi boschi, e arriva fino al mare della Planargia, le cui strade sono punteggiate da vigneti e uliveti, ha vissuto i suoi giorni più drammatici degli ultimi decenni. Eppure, a pochi giorni dalla grande paura, è già in piedi a lavorare per reagire a una devastazione ambientale e paesaggistica, che è già anche economica. La Sardegna ha tirato fuori il suo volto più bello, la "sa paradura", l'aiuto solidale, con camion e trattori che fanno la spola dal resto dell'isola per trasportare mangime e foraggio destinato ai pastori dei paesi del Montiferru, che stanno dando il primo e concreto aiuto. Questo grande lavoro serve innanzitutto a testimoniare lo spirito indomito di quelle popolazioni e di quegli amministratori locali, oltre allo spirito di solidarietà e fratellanza che contraddistingue i sardi nei momenti di grande difficoltà, ma ovviamente non è sufficiente. Le parole di vicinanza, le visite istituzionali e le raccolte di fondi sono a loro volta importanti, ma lo Stato in un momento come questo, già gravato dall'emergenza sanitaria, sociale ed economica che accompagna i territori più deboli del Paese ormai da mezzo secolo, deve dare risposte immediate. Lo deve fare per l'oggi dal punto di vista dell'assistenza economica ai tanti che hanno perso tutto, e per il domani, avviando un confronto con la Regione finalizzato ad affrontare in maniera strutturale e risolvere la questione del governo del territorio. Serve un capitolo dedicato a questi ristori in puntuale coordinamento con la Regione Sardegna e il sistema degli enti locali. Decine e decine di aziende, già di per sé fragilissime, rischiano di essere definitivamente spazzate via in assenza di un intervento più che immediato. Lo spopolamento delle aree interne va di pari passo con il progressivo abbandono delle campagne. Questo è il motivo primo delle mancate manutenzioni dei boschi e dei pascoli, che favoriscono gli enormi incendi e le devastazioni che tutti abbiamo modo di vedere. Il modello di prevenzione, più che quello dei soccorsi a disastro avvenuto, è entrato in crisi e va fortemente messo in discussione. Va ribaltato l'assunto che sia la spesa pubblica, che oggi definiamo improduttiva perché non produce un reddito diretto, sia da demonizzare. Il governo del territorio e la sua manutenzione producono il bene più prezioso: il mantenimento di un ecosistema locale in cui le famiglie, le imprese e i visitatori occasionali possono vivere in armonia con le condizioni di sicurezza e sostenibilità. ai soccorsi, il capo della Protezione civile ha fatto i complimenti alla Regione Sardegna per la sua capacità di reazione e mobilitazione, ma non può essere negato che sussista un problema di risorse

intervengo per ricordare l'immane tragedia vissuta in questi giorni dalla Regione Sardegna nel territorio prima del nuorese e poi dell'oristanese.

tra Forze armate, Vigili del fuoco, ma soprattutto il Corpo forestale e i volontari che debbo ringraziare per il lavoro svolto e per aver salvato vite umane. Purtroppo il mondo agropastorale è a terra e bisogna intervenire immediatamente. La Regione Sardegna ha chiesto già lo stato di calamità, ma ovviamente non basta: adesso occorre un immediato intervento del Governo per risarcire i privati - tante sono le case bruciate - ma anche gli imprenditori, e per ripristinare i boschi bruciati. Ricordiamo che abbiamo perso un ulivo secolare. Occorre investire di più sulla prevenzione, occorre governare il territorio, controllarlo e curarlo, ma occorre soprattutto ripristinare anche il sistema di rilevamento incendi che è cessato che è cessato qualche anno fa. Con questo auspicio abbraccio tutta la comunità sarda colpita e ribadisco la richiesta di un immediato intervento del Governo.

Vogliamo esprimere estrema solidarietà e attenzione al popolo sardo e a coloro che sono intervenuti in soccorso per mettere fine ai roghi che hanno devastato la bella terra sarda. Ci preoccupa la situazione trovo corretto quanto dichiarato dal senatore Cucca: la concomitanza troppo spesso ci porta a vedere la mano dell'uomo dietro a queste condizioni. Rivolgo allora l'appello al Governo di intervenire sul quadro normativo affinché ancora una volta siano presi provvedimenti più severi nei confronti di coloro che si rendono attori di atti atti incendiari che poi devastano il territorio. Esprimo altresì gratitudine per i soccorritori, per i Vigili del fuoco e coloro che si sono attivati in questa circostanza. Vi è certamente disponibilità e volontà da parte del Gruppo parlamentare della Lega per qualsiasi iniziativa che il Governo vorrà proporre per andare in soccorso, anche economico, della terra devastata e consentire alla Sardegna di rimettersi in piedi dopo i devastanti incendi.

Signor Presidente, il lavoro che abbiamo svolto in questi giorni è stato molto complesso. Molti sono gli emendamenti esaminati e approvati. Stiamo terminando i nostri lavori; potremo essere pronti per l'incardinamento per le ore 18, quindi chiedo un'altra ora circa di tempo per concludere l'esame del provvedimento in Commissione.

Non intervengo per stigmatizzare l'ennesima umiliazione del Parlamento - ne parleremo in un'altra occasione - ma chiedo a lei, Presidente, di capire

Ora, scontiamo la litigiosità all'interno della maggioranza (cosa evidentissima), i ritardi della maggioranza e l'ostruzionismo che la maggioranza fa a sé stessa, però non vogliamo esserne vittime. Chiediamo al Governo o a qualcuno della maggioranza che ci spieghi qual è l'intendimento rispetto a oggi, a domani e a venerdì. Tutti noi abbiamo i nostri impegni, abbiamo delle conferenze stampa, delle riunioni

anzi, è arrivato il Ministro - quali sono i tempi, in modo che ci possiamo semplicemente organizzare. È una questione banalmente organizzativa, ma per noi è importante. Sul merito politico avremo altre occasioni in cui confrontarci. Quindi, o ce lo spiega Ministro, ma in maniera dettagliata e attendibile, oppure è meglio convocare una Conferenza dei Capigruppo e decidere come vogliamo procedere. Questo a tutela di tutti, ma anche dell'unica minoranza e dell'unica opposizione in Parlamento. Grazie, senatore Ciriani. Abbiamo ascoltato la richiesta del senatore Parrini di iniziare l'incardinamento alle ore 18 e così intendo procedere. A seguire ci sarà la discussione generale

colleghi, comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale

Signor Presidente, mi dispiace doverle comunicare che non siamo riusciti a terminare i lavori di esame del decreto-legge reclutamento.

il 14 luglio l'ISPRA ha presentato il rapporto sul consumo di suolo per il 2021. Era il giorno in cui l'Europa era flagellata da intense piogge rilevatesi catastrofiche proprio a causa del consumo di suolo. Ne parlo poi oggi, nel mentre disastrosi *flash flood* stanno colpendo la Valtellina e il comasco, Chiavenna, Blevio, Cernobbio con le sue vie trasformate in torrenti furiosi. Dice il rapporto il consumo di suolo, il degrado del territorio e la perdita delle funzioni ecosistemiche continuano a un ritmo insostenibile e, nel 2020, nonostante il *lockdown*, 57 chilometri quadrati di aree agricole e naturali sono state sostituite da nuovi cantieri, edifici e infrastrutture, più di 15 ettari al giorno, un campo di calcio all'ora, due metri quadrati al secondo. Le conseguenze sono anche economiche, e i costi nascosti che l'Italia potrebbe essere costretta a sostenere a causa della perdita dei servizi ecosistemici dovuti al consumo di suolo tra il 2012 e il 2013 sono compresi tra 81 e 99 miliardi di euro, in pratica la metà del *recovery fund*. Nemmeno i rischi idraulici e sismici frenano la cementificazione. Nelle aree a pericolosità idraulica elevata supera il 6 per cento e il 7 per cento in quelle ad elevata pericolosità sismica. I dati evidenziano criticità a livello urbano e periurbano: 2.300 ettari consumati all'interno delle città e nelle aree produttive. Di conseguenza, le città sono sempre più calde e con temperature estive più alte da due a sei gradi centigradi rispetto alle aree limitrofe. sconcertante la crescita di superfici artificiali, anche in presenza di stabilizzazione o decrescita dei residenti. Il suolo consumato *pro capite*, quindi, aumenta, passando da 357 a 359 metri quadrati per abitante. Erano 160 negli anni Cinquanta. consumo di suolo significa perdita di biodiversità, declino del paesaggio, ma anche aumento di superficie impermeabile, così le acque piovane prendono a scorrere anche impetuosamente esondando. Dai dati CNR-IRPI nel 2019 ci sono stati 23 alluvioni, 12 morti, 19 feriti e 3.000 evacuati. Intanto, in Senato recitiamo il *de profundis* alla proposta di legge per il contrasto al consumo di suolo.

si sono convenzionati per svolgere in modo coordinato i servizi sociali e sociosanitari, prevedendo la delega di funzione da parte degli enti sottoscrittori a favore del Comune di Nocera Inferiore. I quattro Comuni, tuttavia, hanno deciso di continuare con le assunzioni precarie con un nuovo bando, anche se ci sono le condizioni per stabilizzare gli operatori, che a partire dal 9 dicembre 2021 avranno maturato i requisiti per la stabilizzazione della

per erogare i quali c'è bisogno di personale assunto a tempo indeterminato. Più volte la Corte di giustizia europea ha sanzionato l'Italia per l'abuso di ricorso continuo al precariato. Le procedure di stabilizzazione per questi operatori nei Comuni indicati, dunque, devono essere avviate al più presto, dando una risposta concreta sia al personale in servizio, sia ai cittadini, per assicurare la continuità dei servizi erogati, soprattutto in questo periodo di emergenza epidemiologica. Si tratta di operatori che da moltissimo tempo, con contratti precari (alcuni superano i si occupano di servizi particolarmente delicati: sono educatori professionali, assistenti sociali, amministrativi, sociologi e psicologi, che assistono quotidianamente le fasce più deboli del nostro territorio. I servizi alla persona, infatti, si fondano *in primis* sulla costruzione di una relazione stabile con soggetti particolarmente fragili che hanno una storia personale complessa. Quindi, non si può assolutamente ripartire periodicamente con operatori diversi. La grande parte degli operatori del Piano di zona è stata assunta a seguito di procedura selettiva il 10 dicembre del 2018 e maturano i tre anni necessari il 9 dicembre 2021. Tutti loro hanno garantito negli ultimi anni - e continuano a farlo - un'azione continua di contrasto alla povertà e presa in carico dei bisogni speciali. Quindi, è un dovere etico e morale che le amministrazioni coinvolte provvedano al reclutamento nei modi indicati dalla legge. Il Consiglio comunale di Nocera Inferiore a fine giugno si è espresso favorevolmente alla stabilizzazione del personale ed alla possibilità di gestire il Piano di zona con un'azienda consortile, mentre il sindaco di Nocera Superiore non era molto d'accordo. In questo continuo ping pong di dichiarazioni e rimpallo di responsabilità anche i sindacati hanno più volte richiesto un incontro, ma non sono mai stati convocati e sono costretti a dichiarare lo stato di agitazione alla prefettura e il Comune di Nocera Inferiore ha confermato un ulteriore bando biennale. Quindi, c'è un rischio concreto che si proceda in questo senso, non avendo cura di assicurare la continuità dei servizi. I sindacati hanno proclamato lo sciopero dei servizi sociali per domani, 29 luglio, nella speranza di avere un confronto proficuo, in modo che si arrivi a una soluzione per i lavoratori coinvolti, ma anche per i cittadini che vengono assistiti quotidianamente. Signor Presidente, nelle ultime settimane sono intervenuto in quest'Aula per denunciare le molteplici azioni contro l'ambiente che si stanno consumando in Sicilia: dall'emergenza rifiuti, che il governo Musumeci intende risolvere bruciandoli, alla pioggia di richieste di autorizzazione per grandi impianti fotovoltaici che rischiano di compromettere il paesaggio e la produzione agroalimentare siciliani; ancora, la volontà di realizzare un inceneritore per fanghi di depurazione nei pressi di Enna, in un comprensorio agricolo di qualità, e gli incendi che stanno devastando l'isola, anche a causa dell'inerzia dell'Amministrazione regionale. Oggi sono qui a segnalare una scellerata norma recentemente esitata dall'Assemblea regionale siciliana: un'anacronistica sanatoria che condona gli immobili abusivi costruiti in aree di pregio paesaggistico e naturalistico, soggette a vincolo, peraltro approvata con un solo voto di scarto. In tal modo si porrà una pietra tombale sulla salvaguardia dell'ecosistema isolano, calpestando la memoria di uomini come Piersanti Mattarella e Bino Li Calsi, che si batterono per tutelarlo, introducendo nel 1978 l'indice di edificabilità sui suoli agricoli. Quanto meno, con un insperato scatto di orgoglio, il legislatore siciliano, durante la stessa seduta, ha bocciato un vergognoso emendamento aggiuntivo al disegno di legge sull'edilizia che intendeva sanare gli immobili costruiti fino al 1983 entro i 150 metri dalla costa. Pochi giorni fa, il collega Ruggiero Quarto ha ricordato le centinaia di vittime e dispersi causate dalle forti piogge in Germania, Belgio e Olanda. Scenari catastrofici come questi devono indurci a riflettere e a compiere scelte adeguate. Un Paese fortemente antropizzato come il nostro ha conosciuto lunghe e generalizzate fasi di abusivismo edilizio, con atti illeciti compiuti anche da enti pubblici che hanno permesso la copertura di corsi d'acqua, la costruzione di edifici in aree soggette a rischio idrogeologico o con vincoli paesaggistici e archeologici. Il condono approvato in Sicilia andrebbe in quella direzione, esponendo la popolazione a gravi rischi e il territorio ai danni causati da un'edilizia incontrollata, preludio all'ennesimo disastro ambientale annunciato. Tutto ciò deve aver fine e la Sicilia non può sottrarsi a questo imperativo. Il Paese che stiamo cercando di disegnare al termine dell'emergenza sanitaria e in linea con le direttive europee deve porsi l'obiettivo della transizione ecologica ed energetica, prevedendo azioni di tutela integrata dell'ambiente e dell'ecosistema. Mi auguro che il grido d'allarme già lanciato da molti contribuisca a bloccare la sanatoria siciliana anche in sede di Consiglio dei ministri, ponendo fine alla stagione dei condoni edilizi. Ce lo impone il tempo in cui viviamo e il futuro che intendiamo costruire per i nostri figli.

dalle enormi proporzioni. Dal 23 luglio scorso, i roghi hanno devastato la zona di Oristano e dell'Ogliastra. Per noi sardi, la piana di Oristano e i monti dell'Ogliastra hanno rappresentato l'agricoltura, l'allevamento, il sostegno economico ed alimentare per tutta l'isola. Oltre 20.000 ettari di territorio, boschi, oliveti e campi coltivati sono ridotti in cenere; aziende agricole sono state distrutte e sono rimaste senza acqua senza corrente elettrica. Molti animali sono rimasti uccisi. Capannoni e fienili con le scorte di foraggio e altre strutture e mezzi sono stati bruciati. Molte case sono state danneggiate. Le attività delle dieci squadre impegnate sono rese particolarmente difficoltose dal forte vento di scirocco, che ha alimentato i roghi, e che più volte ha cambiato direzione minacciando le comunità del Marghine e della Planargia, nonché la strada statale 131 Carlo Felice. Sono stati impegnati otto Canadair, più altri quattro arrivati dalle vicine Francia e Grecia, e tredici elicotteri, in uno sforzo incessante per spegnere il fuoco e salvare il territorio. Le fiamme sono partite dalla zona di Bonarcado e Santu Lussurgiu, ossia nella stessa zona dove ventisette anni fa un incendio scoppiò nel Montiferru. È andato perso un enorme lavoro di rimboschimento e bonifica, attivato dopo tale incendio. Anche in Ogliastra i danni sono rilevanti, nonostante l'intervento quasi immediato della Protezione civile. Sono vicina al vice sindaco di Arzana, impegnato anche con la Protezione civile, giorno e notte, per mettere in salvo tutto ciò che è stato possibile e per tutelare il suo territorio. Ma lui stesso asserisce che l'unico elicottero disponibile, che stava nella vicina Lanusei, nel momento dell'incendio era impegnato ad Oristano in aiuto a quei territori. In Ogliastra non è sufficiente un presidio, ma sarebbe utile un Canadair da tenere in aeroporto di Tortolì in misura preventiva, in modo che per necessità gli interventi possano essere tempestivi. È necessario che la macchina regionale potenzi uomini e mezzi, aerei e terrestri, e disponga una formazione continua del personale, uomini e donne, giovani prestanti utili per svolgere un lavoro duro, ma delicato nello stesso tempo. L'ambiente deve essere difeso da mezzi di avanzata tecnologia, da personale formato assunto a tempo indeterminato e sempre presente per custodire il nostro splendido territorio. la mia solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite e il sostegno affinché le Regioni e il Governo si impegnino al più presto per chi ha perso tutto. È recente la notizia che il ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, in stretto contatto con la Protezione civile, predisporre tutti gli interventi necessari alle aree colpite con eventuali norme e relative coperture finanziarie. Sono in corso interlocuzioni con la Regione Sardegna per valutare l'adozione di misure emergenziali di ripristino. *(Applausi)*.

2025 dopodiché non mi resta che rassegnare le dimissioni da senatore della Repubblica. Non ho altra scelta. Soltanto un paio di mesi fa, a maggio 2021, Torino e, dunque, l'Italia, ricevevano un attestato di fiducia dallo sport mondiale.

Un risultato portato a casa anche dopo l'approvazione da parte del Senato di una serie di mozioni da parte di tutte le forze politiche che tenevano conto delle richieste di tutti i Gruppi e dopo le parole di supporto della sottosegretaria Valentina Vezzali che, partecipando alla cerimonia di assegnazione dei giochi, sottolineava l'importanza dell'evento per il nostro Paese, per lo sport italiano e per il rilancio a livello internazionale della città di Torino. Mi chiedo allora cosa sia potuto accadere per passare da quello che sembrava ormai essere un traguardo certo ad un'ipotesi in bilico che, se non confermata nel giro di pochi giorni, rischia di diventare non solo un'opportunità perduta, ma anche una pessima figura nei confronti della FISU e del resto del mondo. Non si può andare oltre il 31 luglio per validare la scelta del capoluogo piemontese e il finanziamento necessario per realizzare le prossime Universiadi. Esiste altresì un tempo entro il quale occorre salvaguardare il nostro Paese dall'essere percepito come inaffidabile, indeciso e poco credibile. Quel tempo è adesso. Si tratterebbe di un'etichetta che vanificherebbe tutti gli sforzi, la professionalità e le competenze messe in campo in questi mesi, spegnendo al contempo l'entusiasmo di quanti fino ad oggi ci hanno creduto. Mi appello dunque alla serietà e alla concretezza del presidente del Consiglio Draghi affinché non vengano tradite le aspettative di tanti si faccia il possibile per salvare l'Italia da una reputazione internazionale che non rispecchia di certo la nostra storia, la nostra indole e la nostra visione del futuro. **Atti e documenti,